Signor Presidente, colleghi, prima di iniziare il mio intervento vorrei fare una premessa. Parlo da quest'Aula a nome del Movimento 5 Stelle, ma guardando fuori, rivolgendomi al Paese, ai cittadini che stanno al di fuori di quest'Aula. L'Assemblea del Senato esprimerà oggi il suo primo voto su un provvedimento importante, il "decreto Alitalia", che riguarda migliaia di cittadini: ne avremmo voluti affrontare molti altri di decreti importanti, per sostenere famiglie e imprese italiane e, invece, ci troviamo davanti una legislatura che nasce già morta. Non ho alcuna intenzione di perdermi in polemiche: credo siano francamente inutili. Credo sia stato detto tutto; credo che ogni singolo italiano abbia perfettamente compreso ciò che è accaduto in Italia in queste settimane. Nelle recenti elezioni del 4 marzo, 11 milioni di persone hanno sostenuto il Movimento 5 Stelle, che con fatica, ma senso di responsabilità, ha scelto di sedersi ad un tavolo. Mentre l'*establishment* ci tacciava come una forza eversiva, noi abbiamo aperto un dialogo, ci siamo confrontati con un'altra forza politica e abbiamo proposto la realizzazione di un contratto di governo, che contenesse le richieste del popolo italiano. Che piaccia o no, abbiamo riacceso un barlume di speranza per questo Paese; abbiamo ricordato a tutti che la democrazia non è morta; abbiamo ricordato che c'è un'altra via percorribile; ma soprattutto, abbiamo ricordato che esiste un Paese in carne ed ossa, che esistono pensionati colpiti dalla Fornero, 10 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà e migliaia di imprese affogate dall'altissima pressione fiscale. Abbiamo ricordato che le famiglie italiane non sono né numeri né matrici, al contrario di quel che invece ha detto il commissario europeo al bilancio, Günther Oettinger: «I mercati insegneranno agli italiani come votare». Ma ci rendiamo conto? Oettinger si sbaglia: saranno gli italiani ad insegnare a lui il reale valore della democrazia. Questi sono toni intimidatori, come lo sono stati anche quelli di alcuni quotidiani internazionali che, negli ultimi giorni, ci hanno dato degli scrocconi; periodici che ci hanno preso in giro diffondendo l'immagine di un BOT italiano da 5 euro con la foto epica di Marco Tardelli dei mondiali vignette che ritraevano Luigi Di Maio e Matteo Salvini come due malattie che si avventano sul corpo dell'Italia. Quanto ancora possiamo accettare tutto questo? Noi no, non possiamo più accettarlo, ma purtroppo qualcuno lo ha fatto. Come è infatti possibile che un Presidente della Repubblica esprima un giudizio che non riguarda in alcun modo il livello di di un possibile Ministro, bensì il suo pensiero e le sue idee... Ci sono dei limiti costituzionali e non possiamo travalicarli. Presidente: nessuno in questa sede vuole contestare le prerogative costituzionalmente garantite del Capo dello Stato. In quest'Aula forse nessun'altra forza politica come il Movimento 5 Stelle ha lottato per difendere la Carta costituzionale. Ma permettetemi di dire che è inaccettabile porre un veto sulle posizioni e sulle idee di un Ministro, le quali, per logica, rappresentano l'indirizzo politico del Governo e che, a loro volta, rappresentano dunque la volontà di più della metà degli italiani che si è espressa nel voto Non si può pensare di prendere la volontà popolare, metterla da parte e tirare dritti, senza porsi immediatamente e minimamente il problema. Ciò anche perché un tale comportamento può determinare un rischio, ossia che i cittadini si allontanino ancora di più dalla vita politica, disertando persino le urne. L'Italia è tra i primi contribuenti dell'Unione europea e tra i Paesi fondatori dell'Unione europea. Abbiamo sempre onorato i nostri impegni e rispettato i parametri comunitari, a differenza di molti altri *partner* europei che predicavano austerità ai sottoscritti mentre silenziosamente questa austerità la violavano. L'Italia è un Paese che merita rispetto: il suo popolo, il popolo italiano, merita rispetto. merita, Presidente, di poter incidere, perché lo prevede la Costituzione, nel processo politico esercitando il suo diritto di voto. E tutto questo non è accaduto. Anzi, peggio ancora: è accaduto quando il 4 marzo gli italiani hanno alzato la testa con il loro voto, ma sono stati ignorati. Allo stesso tempo, è stato avallato il principio secondo cui è qualcun altro che decide per noi, qualcuno che siede in qualche ufficio a Bruxelles, che passa le ore al telefono con Berlino e che oggi elogia la nascita di un Governo fantasma, sottolineo: un Governo fantasma. Un Governo che non esiste e che forse avremo nelle prossime ore in quest'Aula, un Governo che non esiste signor Presidente, senza una fiducia, senza un perché, senza un'identità, privo di temi e privo di soluzioni. Qui è stato fatto fuori un possibile Governo con una maggioranza solida per mettere dentro un altro Governo che una maggioranza non ce l'ha: ma ci rendiamo conto di che cosa è accaduto in queste ore e in questi giorni in Italia? Un fatto che non ha precedenti nella storia della Repubblica italiana. *(Applausi Ma dov'è la logica di tutto questo? Con che faccia si presenterà il nuovo Esecutivo di fronte a questo Parlamento se nessuno - e sottolineo nessuno - dei Gruppi parlamentari qui presenti ha annunciato che lo sosterrà? Non ci sarà un Gruppo parlamentare che depositerà una mozione di fiducia nei confronti di un Governo. e FdI).* Diventeremo, se dovesse accadere, lo zimbello mondiale e questo non deve accadere, Presidente. Noi, oltre al decreto Alitalia, volevamo fare molto altro: volevamo abolire la legge Fornero, volevamo detassare le imprese italiane per rilanciare la crescita, volevamo introdurre il reddito di cittadinanza che aiutasse chi, magari a cinquant'anni, perde il lavoro e non riesce a reinserirsi immediatamente. Noi volevamo introdurre misure a tutela dell'ambiente, volevamo fare una legge sul conflitto di interessi, che la sinistra in trent'anni non ha mai fatto. Noi volevamo fare una legge contro la corruzione, aiutare i disabili, individuare un piano serio per il Sud volevamo anche rivedere i trattati comunitari che danneggiano la nostra economia e i nostri agricoltori. Volevamo fare tutto questo e non ce lo hanno permesso. Ma se qualcuno, signor Presidente, Presidente, crede che ora ce ne staremo in silenzio, si sbaglia di grosso. Non illudetevi: il Movimento 5 Stelle non molla. Ripeto: il Movimento 5 Stelle non molla, anzi ci state rafforzando ogni giorno di più.

E dobbiamo, giustamente e finalmente, dopo quanto è accaduto, segnare il riscatto di milioni e milioni di italiani. *(Applausi

vorrei far notare ai colleghi che l'Italia, come ha detto giustamente il Capogruppo del Movimento 5 Stelle che mi ha preceduto, merita rispetto, ma non c'è qualcuno in quest'Aula che ha il monopolio della rivendicazione del rispetto. Tutti noi vogliamo rispetto, soprattutto davanti ad affermazioni

perché davanti alla stupidità, all'arroganza, all'autolesionismo, siamo tutti italiani dalla stessa parte. All'onorevole senatore che mi ha preceduto alla stampa internazionale. Per favore, evitiamo di scandalizzarci. La critica a volte dà fastidio, soprattutto quando la si riceve, ma io non ho visto eguale indignazione da parte del Movimento 5 Stelle quando i Governi di Berlusconi, prima, e di Renzi e Gentiloni Silveri, dopo, sono stati attaccati con eguale arroganza dalla stampa internazionale. Silenzio totale. E forse, colleghi, c'è stato anche qualcuno che ha approfittato della lettura di questi giornali internazionali per operare, all'interno del Paese, al fine di delegittimare i Governi - fossero essi di centrodestra o di centrosinistra - che si sono democraticamente susseguiti alla guida del nostro Paese. Qui, colleghi, non siamo all'anno zero. Lo dico perché c'è una rappresentazione di comodo di tutto quello che sta capitando nelle ultime ore in Italia, come se fossimo all'anno zero della democrazia: secondo

e c'è un raggruppamento - una coalizione - che ha avuto la maggioranza relativa. Tuttavia, quello che non era stato detto alcun italiano era che questa coalizione fosse virtuale e che il giorno dopo un pezzo di essa si sarebbe staccato per fare un'alleanza con coloro con cui, in campagna

Mi sembra di essere in un asilo infantile. Dopo trentacinque anni si figuri se ho il problema che qualcuno mi interrompe. Dunque, nessuno ha vinto le elezioni probabilmente va detto agli italiani che questo patto che ci è stato annunciato come il Governo del Paese non era voluto da almeno uno dei due contraenti, che si è preso gioco dell'altro, portandolo

Vi esprimo solidarietà, cari colleghi, perché capisco che essere presi in giro dà fastidio, ma questo è quello che è capitato ed è sotto gli occhi di tutti gli italiani. *(Applausi Infine, esiste la Carta costituzionale. Quello che valeva per tutti i Governi della Repubblica nell'atto della nomina dei Ministri non poteva non valere anche per questo. E se voi difendete la Costituzione, con la tensione morale che avete enunciato, dovete difenderla tutta, non a piacimento e a intermittenza, a seconda dei vostri comodi. Cari colleghi, qui non c'è *in fieri* alcun Governo che espropria. Semmai, c'è un Governo che, per la correttezza istituzionale, viene istituito per evitare che il Governo passato possa gestire, perché frutto di un equilibrio politico diverso, il processo elettorale. sarà semmai un Governo di garanzia, per dare agli italiani la parola che voi richiedete, a dimostrazione del cumulo di contraddizioni che sono state portate anche oggi all'Assemblea del Senato.

Onorevole Presidente, colleghi, la Costituzione è ciò che ci unisce, al di là delle ragionevoli divergenze di indirizzo politico e di idee, appartiene a tutti noi e tutti noi abbiamo il dovere di difenderla, quando essa viene tradita nel suo significato più profondo. In queste ore la nostra Costituzione è minacciata da comportamenti, gesti e intenzioni, che minano le fondamenta della nostra Repubblica. Vi invito, cari colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega, a fare un passo indietro, perché temo che voi non abbiate chiare fino in fondo le drammatiche conseguenze delle vostre azioni.

Sì, ma nessuno ha il diritto di trascinarlo in *bagarre* che nulla hanno a che fare con la tradizione repubblicana. Vorrei dire che in queste ore, per fortuna, stiamo assistendo a una larghissima e diffusa manifestazione di affetto e di fiducia nei suoi confronti e noi di Liberi e uguali ci uniamo convintamente a quelle donne e a quegli uomini di cui siamo fieri e che ringraziamo. Detto questo, sulla situazione politica, come membri di questa Assemblea saremo chiamati a dare dignità parlamentare al dibattito, che si è svolto fino ad ora attraverso roboanti dichiarazioni mediatiche da parte di alcuni esponenti politici in quella circostanza, ciascuno dovrà pubblicamente assumersi le responsabilità delle proprie azioni di queste settimane.

poi fingendo per settimane di perseguire l'intento di formare un Governo politico. Così facendo hanno esposto le istituzioni, l'Italia e tutti i cittadini a pesantissime e pericolosissime sollecitazioni internazionali. Diciamolo chiaramente: vi siete presentati agli elettori forti di due programmi irrealizzabili, in contrapposizione. Poi siete giunti a un accordo al grido di: «Contano i temi e non le persone, i contenuti e non i nomi, le cose da fare e non le poltrone!». Poi, proprio su un nome avete deciso, irresponsabilmente, di non dare avvio a questa legislatura e di lasciare il Paese senza un Governo politico, che pure avete reclamato per settimane, con il basso calcolo di guadagnare qualche consenso in più. Voglio essere chiaro: nel vostro programma - chiamarlo contratto è un'ennesima truffa - c'è un'idea di democrazia che non ci piace, c'è la volontà di fare ulteriori discriminazioni tra gli abitanti del nostro Paese, l'idea che l'Italia sia più sicura armando le persone, che i ricchi debbano pagare le stesse tasse dei poveri e che, comunque, tutto si risolverà cacciando qualche migliaio di stranieri.

la lotta alla precarietà, il contrasto alle diseguaglianze, la sanità pubblica, il superamento della legge Fornero, il rilancio del Mezzogiorno, un piano verde di investimenti pubblici, i temi dell'ambiente, della sicurezza, della giustizia e i diritti civili e di cittadinanza. Voi avete scelto altro: avete scelto di esporre il Paese e i cittadini a grandi rischi (e lo vediamo in queste ore) per il vostro tornaconto. Le urla e gli attacchi di queste ore sono pericolosi; state aizzando i vostri sostenitori contro le istituzioni, contro gli uomini e le donne che le rappresentano. Rappresentare i cittadini è, prima che un grande onore, un'enorme responsabilità; lo dico da uomo che per tutta la vita, con ruoli diversi, ha servito orgogliosamente le istituzioni e che oggi in quest'Aula non intende concedere nulla a chi le ingiuria. In gioco c'è molto più che la contesa politica, qualche consenso in più alle prossime elezioni o una maggiore copertura mediatica nei tg della sera; in gioco c'è molto di più che opposte visioni del futuro dell'Italia. Se consentiamo alla dialettica politica di tracimare in espressioni violente ed eversive, se non ci sentiamo tutti a disagio davanti a certi gesti, allora è la stessa tenuta della nostra comunità che è davvero a rischio. Ciascuna forza politica ha il dovere di prendere le distanze da tali comportamenti, di condannarli e di prendere provvedimenti contro i propri esponenti. È vostro dovere assumervi la responsabilità di chi è chiamato a guidare una comunità politica. Ed è nei passaggi più delicati che si vede la differenza tra chi pensa solo alla convenienza a breve termine e chi ha a cuore il Paese che dice di voler difendere. Pertanto, abbiate il coraggio di porre dei limiti ai comportamenti vostri, dei vostri compagni di partito e dei vostri sostenitori. Per nascondere i vostri errori e i vostri calcoli state fomentando un odio che può travolgere le fondamenta stesse della nostra comunità. Noi di Liberi e Uguali non staremo a guardare. Non possiamo certo, come voi, accettare che il commissario europeo al bilancio ci dica che i mercati ci insegneranno a votare. Ma, allo stesso tempo, crediamo che non esista altro orizzonte se non quello dell'Europa, diversa, radicalmente diversa da quella di oggi. Noi non siamo nazionalisti, non vogliamo uscire dall'euro, non crediamo che la soluzione sia di tornare indietro; rivendichiamo però le possibilità di uno spazio di critica che costruisca finalmente un'Europa un'Europa politica dei diritti sociali e civili, capace di superare, una volta e per sempre, i meccanismi dell'austerità e della speculazione finanziaria. Noi lanceremo, nelle prossime ore, un'iniziativa politica forte, sulla quale ci auguriamo convergano le forze civiche del nostro Paese. Noi spiegheremo ai milioni di cittadini che guardano con preoccupazione alla vostra irresponsabilità che, con le vostre azioni, state mettendo a rischio la qualità della nostra democrazia, la stabilità dell'Italia, la tenuta dell'economia, i risparmi delle famiglie, il credito alle imprese. Voi state aprendo la strada a una crisi ben più forte e profonda di quanto si riesca a immaginare. State ipotecando il presente e il futuro della nostra nazione.

nei giorni scorsi, dall'inizio di questa legislatura così zoppicante, che ha visto sostanzialmente ottantacinque giorni di *impasse* e di stallo. Perché dico che il concetto di sovranità viene anche oggi sacrificato? Lo è,

come si fa a insegnare a qualsiasi popolo quale sia il voto giusto? Troviamo in queste parole una minaccia alla sovranità nazionale, un attacco alle fondamenta della democrazia, e non ho visto alcun alcun rappresentante delle istituzioni italiane inalberarsi e chiedere conto di queste parole. Allo stesso modo, al di là dell'intervento di Tusk, non abbiamo visto il presidente Juncker chiedere una rettifica né intervenire. Tutto questo rappresenta una minaccia per tutti, per la democrazia e per la sovranità. Non sfuggirà a nessuno, né qui né fuori da questa Assemblea, che dal 4 marzo ci troviamo in uno stato, come dicevo, di *impasse* in quella che era inizialmente una crisi politica, una crisi del sistema elettorale, perché abbiamo votato con una legge che Fratelli d'Italia non ha condiviso e che ha gettato il Paese nel caos; dalla crisi politica e del sistema elettorale siamo passati a una crisi istituzionale. Si chiama crisi istituzionale quella che neanche l'intervento del Capo dello Stato riesce a risolvere, e così è avvenuto. Non si è trovata una soluzione con i due mandati esplorativi asimmetrici, e noi sottolineiamo e continuiamo a ripetere che si sarebbe dovuto dare un incarico alla coalizione di centrodestra, nella figura di Matteo Salvini, che aveva comunque ottenuto un consenso popolare che superava il 37 di ottantacinque giorni, siamo ancora a ripetere la stessa domanda: perché non è stata esperita questa strada quantomeno ragionevole?

la fiducia? Lo vedremo. La domanda che continuiamo a fare è perché non è stata esperita e presa in considerazione questa ragionevole via. E perché dico ragionevole? Perché nel 2013 alla coalizione di centrosinistra, che aveva raggiunto una percentuale inferiore che non arrivava al 30

sono andata a leggere con molta attenzione e curiosità non già le tesi di chi, come noi, sosteneva questo, ma di chi respingeva al mittente quanto detto. Ho letto con molta attenzione le tesi di fini costituzionalisti. Non faccio nomi, ma cito testualmente

quando uno vuole parlare delle prerogative del Capo dello Stato non lo può fare in questa sede; ci sono le sedi opportune

della situazione politica. Quando, però, si parla di Presidente della Repubblica, se si critica l'operato del Presidente della Repubblica, lei sa benissimo che c'è un *iter* particolare

regole prevedono che vi siano degli organismi che non sono stati nominati, lo so bene: quindi, anche volendo, non se ne potrebbe parlare. Io sto citando il pensiero di un costituzionalista tratto da un articolo di giornale: questo lo potrò dire in quest'Aula, se l'articolo è stato pubblicato! Il costituzionalista ci parla di sovranità nazionale difesa, quando si è fermata «un'azione politica» - voglio semplicemente finire di leggere - «che puntava a rompere gli impegni europei, che l'Italia ha assunto da cinquant'anni e che è tenuta a rispettare in base all'articolo 11 della Costituzione» - Benissimo! - «La nomina del professor Savona, persona sicuramente competente Allora le tolgo la parola! D'accordo? Se lei non la smette io sono costretta a toglierle la parola! Non stiamo qui rifacendo tutto l'*iter* della formazione di un Governo che purtroppo non c'è stato! D'accordo? SANTANGELO *(M5S)*. E falla

raccolta di firme, una petizione *online* e un appello in difesa della democrazia attraverso un concetto a caro a noi e alla nostra storia, che è l'elezione diretta del Capo dello Stato. Questa è la nostra iniziativa. Concludo dicendo che la prova della democrazia non è se un popolo vota, ma se un popolo governa: questo, dal 4 marzo non è stato possibile realizzarlo!

Signor Presidente, autorevoli colleghi, il presidente Toninelli ha esordito con la considerazione che oggi, finalmente, quest'Aula, il Parlamento, comincia a lavorare su votazioni e discussioni che riguardano l'Italia, il nostro Paese, nello specifico l'Alitalia. Quello che ha omesso di dire, che però dirò io con chiarezza, è perché a questo Parlamento non è stato permesso di lavorare in questi perché le forze che noi abbiamo riconosciuto essere uscite vincitrici dalla tornata elettorale il 4 marzo non sono state in grado o, meglio, non hanno voluto fare un Governo per questo Paese! Non hanno voluto dare un Governo

ha ricevuto una richiesta molto precisa, solo da parte del Partito Democratico: di dare subito le dimissioni. Mi auguro che tutte le altre forze politiche, che oggi fanno finta di contestarlo, abbiano la forza,

Sia la campagna elettorale, sia questi ottantacinque giorni sono stati caratterizzati da troppi malintesi, da cose non dette, in qualche caso anche da falsità e da brutte e cattive interpretazioni degli eventi. Le falsità sono evidenti nei programmi elettorali. La falsità è stata evidente anche nelle aggregazioni elettorali che si sono presentate. Si sono promesse cose che non erano realizzabili: lo si sapeva, tant'è che mai si è spiegato come le cose sarebbero dovuto essere, come i provvedimenti dovevano essere coperti. Ma non è bastato. Non ci si è accontentati del risultato

denso di cose irrealizzabili, di coperture che non esistevano, di provvedimenti che non erano praticabili. Alcuni hanno sottoscritto questo contratto o patto elettorale o di Governo in buona fede. Io credo di sì: credo che alcuni abbiano sottoscritto in buona fede. Altri hanno utilizzato quello strumento per arrivare dove siamo arrivati e dove è che siamo arrivati? Bisogna avere il coraggio di dire la verità e solo perché voi, in maniera irrituale, avete chiesto di parlarne oggi che c'è un altro ordine del giorno, lo facciamo oggi, altrimenti lo avremmo fatto nel Paese. Noi lo faremo

avessero accettato un loro Governo con all'interno un Ministro autorevole, un Vice Segretario della Lega riconosciuto per le sue competenze, che sicuramente aveva le condizioni politiche (sicuramente era stato eletto dagli elettori, cosa che vi dovrebbe suonare abbastanza familiare), oggi saremmo qua a discutere della fiducia al Governo, a discutere dell'impossibilità di realizzare quel contratto, a scoprire quali erano le bugie contenute all'interno del contratto. Ma qualcuno ha teso un tranello. Qualcuno ha voluto giocare sulla pelle degli italiani, prima per aspettare un'elezione regionale, poi per aspettarne un'altra, poi, ha portato la situazione avanti perché si vuole lucrare elettoralmente sulla pelle degli italiani. Le facce di oggi sono chiare: da una parte, c'è la tristezza e la delusione di essere stati presi in giro di quelli che probabilmente erano in buona fede; dall'altra, la soddisfazione di quelli che, da furbi, sono voluti andare avanti su questa strada, pericolosa per il Paese. come è pericoloso quando si parladi *spread* e si dice che alcune forze politiche - nello specifico, l'accusa spesso è verso il Partito Democratico - sono serve dello *spread*. Lo *spread* sono i costi che abbiano sui nostri conti corrente; lo *spread* è il costo che noi, come sistema Paese, dobbiamo pagare per farci pagare quei soldi, lo *spread* è il mutuo della nostra casa; lo *spread* è la nostra

Le bugie erano contenute nei vostri programmi elettorali. Noi abbiamo dimostrato il nostro attaccamento alla comunità nazionale con il nostro programma di Governo e lo abbiamo dimostrato riconoscendo la nostra sconfitta. Lo abbiamo dimostrato aspettando che voi faceste un Governo, che deste delle risposte, che il Paese e il corpo elettorale vi avevano chiesto e che non siete stati in grado e non avete voluto dare a questo Paese.

e portavoce del Movimento 5 Stelle, onorevole Di Maio, e il senatore Salvini hanno chiesto l'istituzione delle Commissioni permanenti di Senato e Camera per cominciare a lavorare. Mi sembra anche questa la solita bugia. Noi, signor Presidente, autorevoli e onorevoli senatori, chiediamo una cosa diversa: un passaggio formale della richiesta di fiducia di questo Governo di servizio - lo definirei un Governo elettorale - per chiedere immediatamente lo scioglimento delle Camere, perché noi sì che vogliamo, a questo punto, andare alle elezioni, noi sì che chiediamo la verifica!

esprimere alcune opinioni che ho condiviso con i colleghi, sentendo parlare chi mi ha preceduto. Innanzitutto, signor Presidente, mi sembra strano che

La sua storia politica ci insegna che cambiando

Colleghi, è sotto gli occhi di tutti che dal 5 marzo ad oggi la Lega con gli alleati di centrodestra e il Movimento 5 Stelle hanno agito responsabilmente nell'interesse del Paese cercando di varare un Governo che potesse iniziare a dare immediatamente delle risposte alle esigenze degli italiani, in un contesto complesso creatosi a seguito del responso elettorale.

Il Movimento 5 Stelle ha cercato un contatto con il Partito Democratico in modo da formare un Governo, ottenendone un rifiuto, in quanto era indisponibile a sedersi ad un tavolo a trattare con i colleghi pentastellati. Poi non diteci che vi abbiamo fatto perdere tempo: abbiamo aspettato per giorni la vostra riunione di partito, perché dovevate decidere di che morte dovevate morire! La Lega ha chiesto, ottenendo una risposta positiva, ai suoi alleati di fare un passo di lato, in modo da provare a trovare un accordo con il Movimento 5 Stelle per dare un Governo al Paese, sempre più inquieto a causa della situazione di stallo politico istituzionale. Lega e Movimento 5 Stelle, faticosamente e generosamente hanno raggiunto un accordo sul programma di Governo, hanno individuato un candidato *Premier*, trovandosi d'accordo sui criteri per la definizione della squadra che quel programma avrebbe dovuto realizzare. Un programma di Governo equilibrato e in linea con quanto necessario al Paese per ripartire e dare fiducia ai nostri cittadini. Un programma di Governo che ha come punti cardine il rilancio dell'economia, la sicurezza, la giustizia, una scuola più efficiente (dopo la vostra "buona scuola", non ci voleva molto), una diversa gestione dei flussi migratori, una politica internazionale che avrebbe dovuto vedere il nostro Paese protagonista, un *Premier* all'altezza e una squadra di Governo composta da rappresentanti politici e tecnici di alto valore riconosciuti in Italia e all'estero. Il tutto con una maggioranza parlamentare, cosa di non poco conto, disposta a concedere la fiducia al Governo che stava per nascere. Nella giornata di domenica abbiamo appreso le riserve del Presidente della Repubblica su alcuni nomi, anzi, meglio, su un nome, riserve che, a nostro parere, nascondono delle riserve sul programma di Governo, a causa di una errata interpretazione e da pressioni mediatiche esercitate anche dalla stampa estera.

Lega e Movimento 5 Stelle, responsabilmente, hanno quindi preso atto della situazione venutasi a creare e dell'impossibilità di dare seguito alla loro idea di dare al Paese un Governo impegnato alla realizzazione di un programma, frutto di un impegnativo confronto, partito da posizioni diverse e talora molto distanti. Lega e Movimento 5 Stelle si sono rimesse alle prerogative che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica e valuteranno con favore qualsiasi ipotesi che consenta alla volontà dei cittadini di esprimere al più presto un voto che assicuri la governabilità del Paese:

Quanto accaduto in queste ore ci lascia basiti e perplessi, Presidente: l'incarico di formare una squadra di Governo al dottor Cottarelli, sapendo benissimo che il *Premier* incaricato non riuscirà a superare la prova delle Aule parlamentari. Un incarico conferito pochi minuti dopo aver bloccato il nostro Governo, che stava per nascere, e dopo un comunicato che ha dipinto quel progetto di Governo come quello di coloro che volevano uscire dall'euro e affossare il nostro Paese. Sfidiamo chiunque a trovare una sola riga del contratto di Governo in cui si parli di uscita dall'euro: sfidiamo chiunque a trovare una sola riga che porti a pensare a un progetto irresponsabile. In queste lunghe settimane il gruppo di lavoro ha sempre operato per dare un futuro migliore ai nostri giovani e mai per mettere in difficoltà la nostra gente*. (Applausi dai Gruppi a quelli che pagano le tasse, a quelli che ogni mattina hanno la fortuna di poter andare a lavorare, a quelli che purtroppo un lavoro non lo trovano, ai nostri giovani costretti a scappare all'estero, a chi aspetta di andare in pensione dignitosamente e a chi in pensione lo è già; agli imprenditori, sommersi dalle tasse, che falliscono per crediti nei confronti di uno Stato solerte a chiedere il pagamento delle tasse, ma cattivo pagatore dei propri debiti. In queste ore, colleghi, un commissario europeo ha affermato: «I mercati insegneranno agli italiani come votare». Gli italiani non devono prendere lezioni di finta democrazia da nessuno, soprattutto dai vostri amici, che avete appoggiato in tutti questi Il nostro motto è «prima gli italiani» (il vostro non lo so, non lo abbiamo ancora capito) e lo rivendichiamo con orgoglio. Non siamo riusciti a realizzare un Governo ora e questo ci dispiace anche per tutte quelle persone che credevano in noi e che ci fermavano per strada e ci incitavano ad andare avanti. Colleghi, noi siamo ricchi di una cosa: abbiamo la forza delle idee; abbiamo la forza dei nostri senatori e dei nostri deputati, che sono stati eletti dai nostri cittadini; abbiamo la forza di tutti quegli uomini e quelle donne che hanno creduto e credono nel nostro lavoro e siamo pronti a votare domani. Signor Presidente, torniamo a votare domani e vi manderemo ancora a casa!

Francamente non colgo lo spirito - ma mi adeguo - di queste comunicazioni. Ritengo che questa sia una discussione che avrà un senso nel momento in cui un Governo si proporrà a questo Parlamento e noi decideremo, ciascuno per la propria parte (mi sembra che ognuno di noi abbia già anticipato i propri intendimenti), se concedere o no

moltissimo orientati, e mi sembra legittimo, ad essere ascoltati dalle persone che ci guardano da fuori - è la nostra posizione rispetto all'Europa. colleghi, alcuni di voi sono reduci da un tentativo di contratto di Governo, noi abbiamo la forza delle nostre posizioni da sempre: in questo momento l'Europa - una porzione dell'Europa, una porzione di rappresentanza dell'Europa - certamente non ci sta aiutando. È evidente che le dichiarazioni del commissario al bilancio Oettinger costituiscano un'offesa nei confronti del nostro Paese. (*Applausi permettersi di dire all'Italia e agli italiani che saranno i mercati a insegnarci a votare! È altrettanto vero, colleghi, che nemmeno noi possiamo permetterci di lasciare il nostro Paese in una situazione di stallo tale che gli italiani, i nostri primi danti causa, i nostri rappresentati, gli europei, il mondo ci guardino con un atteggiamento sospettoso rispetto alla nostra capacità di trovare una soluzione a questa crisi. Guardate, vorrei essere molto chiara con voi, davvero: noi di Forza Italia sul punto dei veti, delle discriminazioni e delle esclusioni non accettiamo lezioni da nessuno. Quando ci siamo presentati in Europa, Silvio Berlusconi, primo tra i grandi *leader* europei, è stato critico nei confronti dell'*austerity*, critico nei confronti dello strapotere dell'euroburocrazia, critico nei confronti dell'asse Parigi-Berlino, o Merkel-Sarkozy che dir si voglia, pagando sulla propria pelle il prezzo di questo atteggiamento critico. *(Applausi fino in fondo, con esclusioni che non solo la nostra storia, ma la storia del nostro Paese, tutta, ancora deve raccontare. una volta, i primi in Europa a dire che era sbagliato fare la guerra alla Libia. Perché faccio questa considerazione, colleghi? Mentre noi scarichiamo le nostre tensioni su noi stessi e sull'Europa, Macron, che in questo momento sta facendo una conferenza sulla Libia, di fatto prendendo il posto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e tentando di esercitare un potere di influenza su una zona che è sempre stata nostra,

sanzioni economiche alla Russia, che per la prima volta nella storia fanno peggio a chi le infligge che a chi le subisce. *(Applausi dal

è il momento in cui veramente tutta l'Europa, il mondo, gli italiani ci guardano aspettandosi da noi un Governo autorevole. Noi lo diciamo, signor Presidente, senza fare citazioni e senza assumere atteggiamenti critici, ma con con una punta di amarezza nei confronti di quello che è accaduto, in questi ottanta giorni e più, dal 4 marzo. Noi avremmo veramente ritenuto opportuno, logico, oserei dire doveroso, che un incarico venisse attribuito a quel centrodestra che non ha solamente acquisito un consenso degli italiani pari al 37 per cento dei voti, ma il 43

su punti condivisi e inclusivi, a guida centrodestra. Abbiamo proposto l'onorevole Matteo Salvini come Presidente del Consiglio, ma non ci è stato assegnato questo incarico. Signor Presidente, non faccio citazioni, ma rilevo con molta amarezza

suggestioni che sono state in passato usate contro di noi - che abbiamo bisogno di un Governo autorevole: questo è il motivo per cui ci siamo determinati a fare un passo in avanti verso la governabilità. Non è bastato. Qual è la soluzione per noi? La più naturale, quella di ridare la parola a chi, solo, in questo momento ha il diritto di parlare: il popolo, il popolo sovrano. Tornare a elezioni riportando Forza Italia nel cammino di un centrodestra unito che sia in grado di riproporre il nostro programma in dieci punti, che è già stato validato dai nostri elettori, dal Paese, che gli hanno garantito e conferito consenso. Questa, onorevoli colleghi, signor Presidente, è la nostra posizione su di un tema che penso meriti, molto più ampiamente di così, di essere sviscerato. Lo ripeto, mi ricollego ad alcune suggestioni per punti che sono state portate all'attenzione di quest'Assemblea, ma soprattutto dell'esterno di questa Assemblea, degli italiani, di tutti coloro che ci stanno guardando, sollecitando però tutti noi, oltre all'apposizione di problemi e alle critiche reciproche, a trovare presto presto una soluzione. La nostra soluzione è questa, ci crediamo fortemente, non possiamo permetterci di portare alla politica ulteriore discredito. Non possiamo permettere che i nostri elettori siano ulteriormente demotivati a manifestare il loro voto e ad esprimere il loro consenso, comunque configurato. Il 10 giugno si voterà per le elezioni amministrative, lo sappiamo. Dobbiamo motivare fortemente il Paese, per far capire che ora abbiamo bisogno che si esprima nuovamente per dare all'Italia quel Governo forte, autorevole, efficace, capace di risolvere i problemi e le emergenze del Paese che in questo momento, qui, non si è generato. *(Applausi

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi mercoledì 23 maggio, ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente, che prevede l'esame dei decreti-legge sulla cessione dell'Alitalia

sedute uniche, con sospensioni tra la sessione antimeridiana e quella pomeridiana, comunicate solo a titolo indicativo. Pertanto, le sedute di domani e giovedì 31 maggio, con orari dalle ore 9,30 alle ore 20, saranno sospese in linea di massima tra le ore 13,30 e le ore 16.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il decreto-legge al nostro esame modifica in tre punti l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del In particolare, si sposta il termine per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia Società Aerea Italiana SpA dal 30 aprile di codesto anno al 31 ottobre 2018. Si sopprime, inoltre, la previsione secondo cui il finanziamento Si sopprime, inoltre, la previsione secondo cui il finanziamento ad Alitalia sia restituito entro il termine dell'esercizio in corso, prevedendo che i finanziamenti concessi per un totale di 900 milioni di euro siano restituiti entro la scadenza del 15 dicembre 2018. La citata norma, vigente fino all'entrata in vigore del decreto in esame, ossia l'articolo 12, prevede infatti due scadenze differenziate: per la quota di 600 milioni di euro, erogata con decreto-legge n. 50 del 2017, la restituzione è prevista entro il 30 settembre 2018, mentre per la quota di 300 milioni di euro, concessa con decreto- legge n. 148 del 2017, la restituzione è prevista entro il termine dell'esercizio dello stesso anno 2018. Sul piano tecnico, i prestiti in questione, rispettivamente concessi per indilazionabili esigenze gestionali e per evitare l'interruzione del servizio pubblico, sono garantiti dalla prededucibilità e hanno danno un'onerosità pari all'Euribor a sei mesi maggiorato di 1.000 punti base. Il tasso attualmente è pari al 10 per Si segnala che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame afferma che la norma non determina nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né alcun effetto finanziario, atteso che la nuova scadenza del finanziamento ricade nel medesimo esercizio precedentemente individuato. Come rilevato anche dal Servizio del bilancio del Senato, andrebbe comunque verificata l'assenza di effetti finanziari sul fabbisogno derivante dalla proroga, di due mesi e mezzo, della restituzione della quota di 600 milioni di euro del finanziamento. Ciò nella misura in cui si potrebbero determinare maggiori oneri ed esigenze finanziarie dello Stato, che per finanziarsi, potrebbe far ricorso ad emissioni di titoli del debito pubblico, con connessi oneri per interessi. È opportuno soffermarsi sulle alterne e a tratti irresponsabili vicissitudini che hanno caratterizzato, da oltre due lustri, la conduzione delle problematiche che hanno investito, purtroppo, la nostra compagnia di bandiera. È doveroso inoltre rammentare che l'attuale Società Aerea Italiana SpA è giunta all'ingloriosa conclusione di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, da ultimo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano). Con il medesimo decreto è stato nominato il collegio commissariale della società, in un numero di tre componenti, di cui uno già facente parte del precedente organo amministrativo. La documentazione posta a corredo del decreto di ammissione alla procedura straordinaria, resa nota solo recentemente, evidenzia una situazione patrimoniale ampiamente deficitaria. I dati aggiornati alla data del 28 febbraio 2017 mostrano una situazione così strutturata: un *deficit* patrimoniale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2447 del codice civile, con capitale proprio al di sotto del minimo di legge, ovvero negativo di 72,8 milioni di euro, dovuto a persistenti perdite economiche conseguite, pari a oltre un miliardo di euro; un manifesto stato di insolvenza derivante da una permanente situazione di squilibrio monetario, con passività correnti, ovvero scadenti entro i dodici mesi, di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di attività correnti disponibili di soli 921 milioni di euro, insufficienti a soddisfare gli impegni assunti; uno squilibrio finanziario strutturale, con una debitoria complessiva di oltre 3,2 miliardi di euro, sbilanciata sul breve termine e indirizzata inspiegabilmente a finanziare, per circa un miliardo di euro, attività finanziarie non produttive, ovvero crediti finanziari e derivati. Sul piano tecnico operativo le cause di questo fallimento annunciato vanno ricercate principalmente nel modello di *business* adottato, il quale ha privilegiato soprattutto voli di breve raggio, con conseguente irragionevole disimpegno progressivo dell'offerta sui collegamenti intercontinentali. Questo ha esposto Alitalia a subire la crescente concorrenza delle compagnie *low cost*, con conseguente caduta graduale della redditività. Le scelte strategiche sono state condizionate in parte dalle esigue risorse investite dai soci di Alitalia, insufficienti a sostenere investimenti durevoli e a favorire strategie commerciali maggiormente redditizie dei voli di lungo raggio. In questa errata visione strategica è stata ridotta progressivamente la flotta degli aerei per i collegamenti extraeuropei e sono stati venduti nel 2014 a Etihad, dopo il suo ingresso nella compagine sociale di Alitalia, persino i diritti di decollo e atterraggio, i cosiddetti *slot*, sull'aeroporto londinese. Su quest'ultima operazione, seppur persistano dubbi sulla convenienza economica dell'operazione in sé, che di fatto ha costretto l'azienda a privarsi di un importante *asset* strategico, permane, a detta dei commissari, la possibilità di poter riacquistare detti diritti allo stesso prezzo di vendita realizzato. Nel corso della gestione ante-commissariamento hanno inciso sulle menzionate perdite economiche sia la sensibile riduzione dei ricavi operativi, in particolare di quelli attinenti ai passeggeri, sia gli elevati costi della flotta, riconducibili principalmente agli extracosti dei contratti di manutenzione e di *leasing*, sia gli alti costi del sistema informatico e degli oneri finanziari, tra cui quelli sui derivati per la copertura del rischio di cambio e delle oscillazioni del rialzo del carburante. Questi ultimi sono risultati tanto esosi quanto pleonastici, in un periodo di continua riduzione dei prezzi del petrolio. A seguito dell'ammissione all'amministrazione straordinaria si è assistito ad un vero e proprio vuoto informativo, che inevitabilmente ha accresciuto il clima di sfiducia degli *stakeholder* e che potrebbe influire sulla stessa procedura di cessione del complesso aziendale tutt'ora in corso. Non risulta infatti redatto ed approvato, ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, il bilancio di esercizio 2016, il quale, come noto, avrebbe dovuto essere deliberato entro il 30 aprile 2017, l'assenza di documentazione contabile in seno alla richiesta di ammissione alla procedura straordinaria. In sede di indagine conoscitiva, infatti, è emerso che non risulterebbero depositate, presso la cancelleria del tribunale, la situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni dalla richiesta di ammissione alla procedura, il deposito della documentazione contabile e la relazione sulle cause. L'assenza di informazioni contabili è stata in parte riscontrata anche in seno alla medesima gestione commissariale, laddove lo stesso comitato di sorveglianza ha confermato la mancata redazione delle relazioni trimestrali *ex* articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999, da presentarsi al Ministero dello sviluppo economico a decorrere dall'inizio della procedura di amministrazione straordinaria. Sempre sul piano informativo, si rileva la non tempestiva comunicazione del Governo italiano alla Commissione europea in merito al prestito concesso, avvenuta solo a gennaio 2018 per l'intera cifra erogata (900 milioni di euro). ha fatto seguito a una serie di denunce che la Commissione europea ha ricevuto nel 2017, nelle quali si sosteneva che il prestito costituiva un aiuto incompatibile con le vigenti norme europee. Il comunicato stampa della Commissione europea del 23 aprile 2018, che riporta le dichiarazioni della commissaria responsabile per la concorrenza, riferisce che è in corso un'indagine approfondita per valutare se il prestito costituisca un aiuto di Stato

articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). In particolare, la Commissione teme che la durata del prestito superi la durata massima di sei mesi prevista dagli orientamenti per i prestiti di salvataggio e nutre dubbi sul fatto che l'aiuto si limiti al minimo necessario. L'entità del finanziamento concesso, infatti, più che sopperire a un momentaneo stato di necessità, sembra concesso per avviare una ristrutturazione senza che sia stato presentato preventivamente il relativo piano di salvataggio.

I dati emersi dalle audizioni hanno comprovato le politiche di risanamento avviate dai commissari, rivolte principalmente a salvaguardare i ricavi operativi e a contenere i costi strettamente di funzionamento. Gli esiti gestionali, però, sono ancora contrastanti. Particolarmente significativi risultano le riduzioni dei costi operativi, così come l'aumento dei ricavi. i risultati finali del periodo maggio-dicembre evidenziano ancora un risultato economico negativo di -168 milioni di euro. Ad aggravare il citato quadro economico, va tenuto presente che l'esaminata situazione economica non ha considerato gli aspetti negativi non ricorrenti, nonché l'incidenza degli oneri finanziari. In funzione di tale possibile prospettiva, la Commissione speciale ha esaminato, discusso e approvato riformulato nel testo 2, alla luce del complesso delle proposte emendative presentate. È sotto gli occhi di tutti che, nel caso in cui non dovessero intervenire soluzioni di carattere straordinario, quali l'accesso di nuovi investitori e/o la partecipazione statale al capitale di Alitalia, sarà inevitabile assistere all'ennesimo fallimento della società, da cui conseguirebbero gravi e incontrollabili problemi occupazionali, sociali ed economici. Diventa pertanto irresistibile, e più che mai attuale, citare la famosa frase del grande Nietzsche: «Il rimedio è stato peggiore del male». *(Applausi

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà. Signor Presidente, è con vero piacere che posso appellarla con questa tale qualifica in quest'Aula, dopo aver lavorato alcuni anni insieme.

Il comma che veniva aggiunto aveva una sua connotazione specifica che era corretta, ma la mia preoccupazione e quella del mio Gruppo era

ovvero una compagnia di bandiera, ma questo dovrebbe fare i conti con i costi e con la possibilità di continuare a gestirla.

si caratterizzi per un'attenzione particolare alle necessità del nostro Paese. Il nostro Paese deve competere sotto il profilo della concorrenza turistica

e sui nostri aeroporti. Vi è una necessità. Ebbene, se vi è una necessità di vendita, dobbiamo fare in modo che, contestualmente, vi sia un apprezzamento del mercato nei confronti di un marchio. Abbiamo una fortuna. Il marchio Alitalia, ancora oggi, nel mondo ha una sua caratterizzazione e una

cioè, la possibilità di insegnare agli altri come gestire la manutenzione degli aerei. un marchio che, quindi, ha un valore ancora oggi. Ciascuno di noi che ha un'esperienza minima di volo anche con altre compagnie,

togliere quella aureola di bravura che caratterizza l'Alitalia e che noi dobbiamo garantire per arrivare

a una compagnia di bandiera. Perché questo si realizzi è necessario un Governo forte, che abbia la capacità di dialogare su queste materie.

anche se si fosse trattato di quello politico appena nominato. Occorre, invece, avere quel minimo di *spatium deliberandi* perché possa realizzarsi al meglio meglio un obiettivo che io interpreto come comune dopo quello che abbiamo detto in Commissione e che qui ha ribadito il relatore. Per questo motivo io voterò a favore del provvedimento.

Signor Presidente, interveniamo oggi in quest'Aula in un clima surreale. Stiamo parlando di un argomento fondamentale per la nostra Nazione ma è chiaro che la nostra testa purtroppo è altrove. Cerchiamo di essere concentrati su un argomento altrettanto importante, ma è evidente che il clima è abbastanza surreale. Mi verrebbe quasi da dire che, anziché parlare di Alitalia, stiamo parlando di "Ah, l'Italia" per quei discorsi che abbiamo fatto fino ad ora. Mi permetto di dire una cosa a lei, signor Presidente, perché lei è la nostra rappresentante ed è stata eletta da noi.

poi ascoltare quello che invece sta accadendo al di fuori di quest'Aula. Ma veniamo al tema di questo decreto-legge. Questo decreto-legge verrà convertito, non so da quale maggioranza. Non sappiamo chi sia seduto in quei banchi e se sia qualche reminiscenza di un che, molto probabilmente, a luglio scomparirà definitivamente dalla memoria degli italiani, oppure magari M5S)*. È chiaro che gran parte dei problemi di cui stiamo discutendo è stato generato proprio da voi. È stato generato anche all'interno del Ministero dove la vice ministro Bellanova ha

completamente depauperato del potere che ci è stato assegnato. È vero anche nel caso Alitalia perché è stato gestito in una maniera che abbiamo contestato. Non siamo mai stati informati su quanto accadeva. È vero per questa vertenza, ma anche per molte altre che sono passate anche per il suo tavolo, Vice Questo noi lo abbiamo sempre detto. Noi abbiamo contestato in passato questo metodo di affrontare le questioni e lo contesteremo anche in fase emendativa chiedendo più informazioni.

Questo è un tema che probabilmente nella prossima legislatura dovremo affrontare e rivedere completamente. Dovremo ripensare completamente a come il Governo italiano e l'Italia gestiscono le crisi d'impresa. Sicuramente non come lo avete fatto voi finora.

Sicuramente non me lo dirà il commissario Oettinger, ma il mio collega e amico, senatore Cioffi, che è un cittadino eletto democraticamente dai cittadini italiani perché il mio voto conta! Grazie

al fine di massimizzare i risultati della liquidazione, garantire i creditori sociali, conservare il patrimonio produttivo dell'impresa e salvaguardare i livelli occupazionali (che è ciò che veramente ci interessa in questo momento).

Siamo davanti a un finanziamento già in corso di 600 milioni di euro, che è stato concesso per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società Alitalia, mentre quello aggiuntivo è volto a garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto ed evitare l'interruzione del servizio pubblico aereo. È questo il motivo per cui il decreto-legge in esame ci interessa e per cui lo voteremo. Sulla sorte di Alitalia è stato fatto molto lavoro, in particolare dagli enti locali (di cui ho seguito moltissimo il lavoro), *in primis* dalla Regione Lazio, dal Comune di Fiumicino e dal Comune di Roma. Vi dovrebbe interessare, cari colleghi, perché anche il Comune di Roma si è occupato della questione Alitalia. Questi enti locali se ne sono occupati per non restare con le mani in mano a guardare cosa succede, ma per cercare di dare un contributo con soluzioni e proposte. Una cosa è certa: si tratta della più grave crisi occupazionale che colpisce il territorio della Regione Lazio tutta l'area romana, con epicentro nel Comune di Fiumicino. Proprio per questo sono state presentate dai nostri enti locali proposte di rilancio della compagnia, chiamando in causa le grandi aziende a partecipazione dello Stato che si occupano di trasporto, di energia e di manutenzione. Oltre al piano precedentemente presentato, si può comunque fare un'analisi approfondita e dare ulteriori contributi. Non è il caso di analizzare solo lo stato di crisi di Alitalia, ma occorre provare a segnalare anche possibili linee di sviluppo per la compagnia che con la proroga offerta dal decreto-legge in Partiamo dall'analisi delle principali cause dei tre *default* successivi che, uno dopo l'altro, in meno di dieci anni hanno colpito l'Alitalia. Per farlo, ci si può soltanto rifare al bilancio 2015, perché è l'ultimo bilancio pubblico depositato. Da quel bilancio di esercizio 2015 si evincono le principali criticità che affliggono Alitalia da tempo immemore e che mai hanno trovato soluzioni serie, reali e concrete; opportuno precisare che il teorema secondo cui Alitalia è una palla al piede per lo Stato italiano che incide da decenni sulle tasche dei contribuenti ha un elevato tasso di qualunquismo misto a populismo. Alitalia è una grande impresa italiana e, come tale, merita ogni sforzo per il suo salvataggio. Sia chiaro a tutti che Alitalia non è una qualunque impresa privata; Alitalia è stata ed è ancora il biglietto da visita del nostro Paese nel mondo e, come ha ben detto il collega Caliendo, ha comunque un valore importante per molti consumatori di ogni continente che ancora oggi scelgono Alitalia malgrado gli eventi accaduti dal 2008 ad oggi. Sono oltre 20 milioni i passeggeri trasportati - sempre secondo i dati 2015 - con una flotta sottodimensionata e disomogenea, ma sono la prova tangibile che ancora c'è fiducia in questa azienda. Appare inoltre inconcepibile che un Paese a vocazione turistica come il nostro possa rimanere senza la propria compagnia di bandiera, considerando l'incidenza della voce turismo sulla nostra bilancia commerciale.

500 milioni per il personale; 400 milioni per costi legati alla manutenzione della flotta; 300 milioni per i costi relativi alle operazioni di scalo, *handling* e diritti aeroportuali; 250 milioni imputabili ai diritti di sorvolo e infine 100 milioni imputabili ai costi per il sistema di prenotazione e vendita dei biglietti. Tra i costi evidenziati, questi numeri che vi ho letto, questi otto elementi di costo, gli unici che per incidenza si trovano ad essere in linea con gli *standard* europei di tutti gli altri Paesi, sono quelli relativi al personale e ai diritti di sorvolo, i diritti aeroportuali. Tutte le altre voci di costo sono palesemente lontane da ogni logica reddituale. Esaminiamo adesso la prima voce, quella più spropositata di tutte, il costo del carburante che incide addirittura sul costo pieno per circa il 20 per cento. Considerando il numero di aerei in flotta, la loro tipologia, i percorsi e le ore volate nell'esercizio relativo all'anno 2015, risulta che Alitalia abbia pagato per il carburante intorno al 20 per cento in più rispetto ai valori di mercato. Altra voce da tenere presente è quella dei costi relativi al *leasing* degli aeromobili. Alitalia ha i peggiori contratti di *leasing* mai negoziati in aviazione moderna e non solo per il rateo mensile riferito al nolo degli aeromobili che è di circa il 15 per cento maggiore della media di mercato, ma anche per condizioni economiche relative alle riserve di manutenzione e alle condizioni di riconsegna che sono assolutamente spropositate, totalmente fuori da ogni logica di mercato e gravano sui conti della compagnia per centinaia di milioni. Se ciò non bastasse, dovete sapere che Alitalia noleggia alcuni aeroplani secondo una formula definita Wet Lease o ACMI che è l'acronimo con cui si definisce un modello di noleggio che comprende, oltre l'aeromobile (*aircraft*) anche l'equipaggio (*crew*), la manutenzione del velivolo (*maintenance*) e l'assicurazione dello stesso (*insurance*). Questa formula di noleggio è assolutamente antieconomica e venne istituita solo per dare la possibilità alle aerolinee di potere far fronte ad eventuali avarie di un aeromobile della propria flotta, sostituendolo per un periodo limitato con un aeromobile operato da altra compagnia soprattutto allo scopo di tutelare la carta dei diritti del passeggero in materia di riprotezione del volo. Alitalia invece, facendo un grave errore, utilizza questa formula di noleggio con Ethiad regional (che altro non è che la compagnia regionale svizzera Darwin) operando tratte che invece potrebbero essere operate in proprio con i componenti della propria flotta con notevoli risparmi. Viene da pensare che forse occorreva aiutare la compagnia svizzera nell'impiego degli aeromobili, nell'interesse esclusivo del socio che altrimenti avrebbe dovuto coprire anche le copiose perdite di Darwin, oltre quelle di Air Berlin. Veniamo ad un'altra voce di spesa sempre piuttosto importante che è quella relativa ai costi della manutenzione degli aeromobili. Alitalia, dal 2008 in poi, inizia un processo di esternalizzazione della manutenzione che è una delle cause primarie dei successivi dissesti dell'aerolinea. Chi di voi frequentava i lavoratori dell'aeroporto - Presidente le chiedo un attimo ancora si ricorderà quali e quanti erano gli *hangar* di manutenzione, quale immenso lavoro si faceva sui motori, sulla componentistica e sulla parte interna degli aerei. Bene, quegli *hangar* di manutenzione non esistono più, sono stati interamente smantellati. È stato fatto un accordo con una compagnia israeliana. Alcuni motori vengono caricati sui cargo e spediti in Israele per essere aggiustati, smantellando non solo tutta la parte degli *hangar* ma anche l'immensa ed infinita competenza dei nostri lavoratori.

sui punti più importanti. Come potremmo, davanti all'ipotesi di approvazione di questo decreto-legge che allunga i tempi, ottenere dei risparmi? Alitalia risparmierebbe circa 150 milioni di euro annui rispetto ai costi di manutenzione, come vi ho detto; verrebbero ad essere reimpiegate migliaia di unità lavorative oggi in cassa integrazione; verrebbero ad essere reimpiegati anche *hangar* e numerose strutture; verrebbe restituita dignità professionale a ingegneri aeronautici, meccanici e professionisti; Alitalia potrebbe vendere a terzi i servizi di manutenzione prodotti in casa; si potrebbe ottimizzare la flotta in relazione alla soglia dimensionale e strategica di questo *network*. Concludo, signor Presidente, nel dire

nel valorizzare le competenze e la qualità professionale che caratterizzano non pochi soggetti all'interno della compagnia. Si pensi ad esempio al ritorno in termini economici e non solo che si potrebbe ottenere nel ricostruire un scuola del volo Alitalia. Certamente, considerata la qualità e la tradizione dei piloti italiani, potrebbe diventare punto di riferimento di molte compagnie nel mondo ad iniziare da quelle cinesi e da quelle dei Paesi emergenti (Arabi compresi) che necessitano costantemente di competenze

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che siamo chiamati oggi a convertire in legge detta misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. In particolare, esso differisce al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento di tali procedure di cessione e proroga al 15 dicembre 2018 la durata del finanziamento a titolo oneroso di 900 milioni di euro, sopprimendo le disposizioni che ne prevedevano ne prevedevano la restituzione entro il termine dell'esercizio. Tale esigenza nasce per ben valutare e ponderare, oltre all'offerta economica e di acquisto, anche la politica industriale sottesa alle stesse offerte. Il lavoro svolto in Commissione speciale al Senato è stato meritorio e valido e per questo ringrazio i colleghi senatori. Si è acquisita la posizione dei tre commissari straordinari, dei tre Ministeri coinvolti e dei sindacati. Colleghi, Presidente, dare il via libera alla conversione del decreto-legge, accettando la proroga sui termini delle procedure di cessione di Alitalia, non significa spingere per una cessione della compagnia di bandiera; si tratta, bensì, di un atto di responsabilità nei confronti dell'azienda e di chi ci lavora, soprattutto alla luce dello stallo politico attuale. serve un rilancio da attuare, consentendo allo Stato di fare tutto il possibile e, in prospettiva, di realizzare una vera e grande compagnia di bandiera, che sia espressione del *made in Italy*, dell'italianità e del genio

una delle più importanti e preziose vetrine internazionali, ricca di storia, di tradizioni, di beni architettonici e culturali che conosciamo tutti, di paesaggi incantevoli, di clima e luoghi invidiabili, che permettono di sfruttare le quattro stagioni favorendo il turismo,

che, decidendo di visitare l'Europa, trovano comodo raggiungere il nostro amato Paese, anche per l'offerta che deriva dalla compagnia stessa. Investire sulle tratte a lungo raggio, che sono quelle più remunerative, non solo permette di rilanciare l'azienda con l'aumento del numero dei passeggeri, ma permette anche di aumentare il PIL del nostro Paese con un maggior numero di visitatori che portano ossigeno alle nostre piccole e medie imprese. Per tale ragione, serve il tempo necessario per la scelta di un *partner* industriale che tuteli gli interessi italiani evitando che l'Alitalia diventi una compagnia regionale di un altro vettore europeo. La flotta dell'Alitalia è troppo incentrata verso il corto-medio raggio, il segmento con più concorrenza, mentre è estremamente debole rispetto ai *competitors* per le rotte intercontinentali, che consentono i margini di maggiore ricavo. ricavo. Il *management*, prima, ed i commissari, poi, hanno ridotto i costi operativi, ma hanno potuto fare ben poco senza investimenti nella flotta a lungo raggio. Occorre avere più tempo per ripensare la politica industriale, unitamente al *partner* commerciale che verrà individuato dal prossimo Governo, avendo di mira il complessivo sistema dei trasporti, senza politiche a compartimenti stagni ovvero misure tampone che si limitino a differire le decisioni. Occorre una visione unitaria e sistematica che consenta di garantire il trasporto come servizio pubblico essenziale, diversificando l'offerta senza mettere in concorrenza inutilmente comparti differenti: penso all'Alta velocità ed al trasporto aereo,

va al Sud, che deve essere al centro del progetto industriale della compagnia aerea, perché esso rappresenta un potenziale turistico fondamentale per il rilancio, non solo del territorio, ma anche e soprattutto dell'intero Paese. La conversione in legge del del decreto-legge che oggi ci accingiamo a varare deve essere un punto di partenza per ridare dignità ed efficienza ad un settore strategico e fondamentale per lo sviluppo futuro del nostro amato Paese e, naturalmente, a tutela della nostra Alitalia.

questo dibattito conferma come il tema della salvezza della nostra compagnia di bandiera e il suo rilancio siano un nostro dovere primario per difendere migliaia di posti di lavoro, anche nelle aziende dell'indotto che offrono servizi in tutti gli scali italiani, da Napoli a Fiumicino, da Milano a Palermo, e il ruolo strategico che il nostro vettore sta svolgendo a casa nostra e nel mondo per chiudere una lunga fase, come hanno iniziato a fare i commissari incaricati, di errori e sprechi. La gestione commissariale ha conseguito risultati apprezzabili sul piano della riduzione dei costi e dell'aumento dei ricavi. Le perdite sono state ridotte rispetto alle gestioni precedenti e si prevede un ulteriore miglioramento durante la stagione estiva senza considerare i risultati operativi raggiunti, che vedono Alitalia da mesi stabilmente tra le prime compagnie del mondo per puntualità. Questi risultati - occorre sottolinearlo sono stati raggiunti senza intaccare il prestito concesso dal Governo. Ciò dimostra che la nostra compagnia può ancora recitare un ruolo fondamentale nel mercato del trasporto aereo, soprattutto per la connettività del nostro Paese.

o partono direttamente per una destinazione internazionale e intercontinentale ce ne sono sessantadue che devono fare almeno uno scalo negli *hub* dei maggiori vettori europei per raggiungere la destinazione finale. Questo dato è fondamentale per capire che il Paese ha bisogno di un vettore nazionale che non sia al servizio di altre compagnie alimentando i loro *hub*, ma colleghi l'Italia con il resto del mondo per favorire il turismo e l'imprenditorialità. La compagnia, anche come motore di sviluppo nazionale, può essere rilanciata mediante il coinvolgimento di nuovi soggetti pubblici e privati, disponibili a investire capitali adeguati nell'attuazione delle linee strategiche individuate durante la gestione commissariale, soprattutto per il rinnovamento della flotta e lo sviluppo delle rotte intercontinentali. Il rilancio può passare anche per un riequilibrio del mercato del trasporto aereo nazionale mediante regole trasparenti, soprattutto in materia di incentivi da parte degli aeroporti ai vettori *low cost* nell'ambito di un più ampio sistema nazionale di trasporti integrato. Vorrei cogliere, per gli ultimi secondi che restano del mio intervento, quest'opportunità per dire che il tema Alitalia si collega al più generale tema della logistica nel nostro Paese. Ci sono grandi novità nella geografia della logistica, che riguardano il Mediterraneo e che interessano direttamente il Mezzogiorno d'Italia e l'Italia. C'è un grande interesse di grandi *player* internazionali; c'è la Cina che sta attuando moltissime attività geostrategiche sul piano della logistica, con attenzione rivolta al Mediterraneo. Noi abbiamo fatto delle cose importanti con i Governi che ci hanno preceduto, ma dobbiamo insistere nel rafforzare l'intelaiatura logistica del nostro Paese,

tutto ciò che può consentire al Mezzogiorno d'Italia e all'Italia di svolgere un ruolo di *hub* nel Mediterraneo. Questa opportunità, signor Presidente, non la dobbiamo perdere. Se questo significa fare alleanze in Europa, che non vuol dire andare con il cappello in mano verso qualcuno, lo dobbiamo fare, perché se non saremo presenti nelle grandi sfide europee e internazionali

Signor Presidente, onorevoli colleghi, da professionista, da uomo d'impresa, sono felice di parlare in questa sede di argomenti concreti qual è l'argomento di Alitalia, un argomento sicuramente drammatico e che da anni attanaglia il nostro Paese e la nostra economia. Dispiace, però, constatare che di questi argomenti e di questa concretezza avremmo avuto tanto bisogno di parlare anticipatamente. Sono ormai tre mesi, signor Presidente, che siamo senza un Governo; sono tre mesi che il nostro Paese aspetta di vedere l'amministrazione agire su problemi veri e concreti - quali, appunto, quello dell'Alitalia - e credo che sia un *record* nella storia repubblicana: nessun politico, nessun amministratore si è presentato come candidato Presidente a chiedere la fiducia in una Camera e precisamente al Senato della Repubblica. Questa è una vera criticità, una drammaticità che stiamo vivendo e alla quale noi tutti dobbiamo saper rispondere con senso di responsabilità. Quindi, eccomi sull'Alitalia: «misure urgenti su Alitalia», come recita il titolo delle note senatoriali su questo decreto-legge. Già qui mi sento di apostrofare il Governo con una critica, perché quando noi professionisti, noi uomini d'impresa, dobbiamo chiedere una proroga per i nostri lavori, già siamo in difetto e quando poi la proroga magari è la seconda, molti di noi verrebbero mandati a casa. Ebbene, qui siamo a chiedere una seconda proroga su un decreto per Alitalia che - ricordo a noi tutti vuole ora spostare al 15 ottobre i termini per l'espletamento della procedura di gara. Ebbene, siccome nessuno di noi è ingenuo, ore saremo qui chiamati a votare su un decreto di proroga al 15 ottobre, quando sappiamo benissimo, anche sulla base delle audizioni che ci sono state, che non c'è nulla di concreto in termini di acquisizioni di Alitalia.

stiamo entrando in una procedura di infrazione. Sappiamo benissimo che la normativa comunitaria concede dei prestiti per il finanziamento delle situazioni di emergenza, ben condizionati: al rimborso entro sei mesi ovvero come alternativa, a un piano di ristrutturazione. Oggi non è prevedibile un rimborso, appunto perché si chiede un rinvio, ma non abbiamo nemmeno la benché minima idea di un piano di ristrutturazione della compagnia. Questi sono i problemi che ci stanno attanagliando. I signori del Governo presenti oggi in Aula dovrebbero rispondere del perché siamo arrivati a questo punto. Il Governo Gentiloni Silveri dovrebbe rispondere al popolo italiano del perché questa compagnia aerea da oltre un anno in questa situazione. Addirittura, per chi non lo sapesse, la precedente amministrazione è sotto inchiesta presso la procura di Civitavecchia per bancarotta fraudolenta. La scorsa settimana gli uffici dell'Alitalia sono stati visitati dai militi della Guardia di finanza per i gravi dubbi che stanno attanagliando la procura.

a noi tutti come possiamo interrogarci su questo tema, al di là del voto che esprimeremo. Di certo

dove vuole andare Alitalia. Vorremmo capire meglio cosa è successo quando sono stati ceduti in modo piuttosto controverso - per non dire preoccupante, secondo la procura della Repubblica - gli *slot* a quell'Etihad che era parte della nostra compagnia. Tali *slot* sono stati ceduti a un valore che sembra essere nettamente inferiore a quello reale. Quindi, si è svenduto un patrimonio di Alitalia e, peraltro, non si è neppure attivata la clausola che avrebbe permesso e permetterebbe di rientrare in possesso di questi beni. di criticità importanti e responsabilità ancora più gravi del Governo su questo tema. Pertanto, ora non sappiamo dove dovremo andare. in Commissione abbiamo sentito che le prospettive che potrebbero delinearsi sono quelle delle rotte internazionali, per le quali però servirebbero degli ingenti investimenti. Si parla di oltre un miliardo di euro già dal primo anno;

esprimendo una seria preoccupazione al riguardo. Sarà poi il nostro Capogruppo a esprimere la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia su questa proroga e sul decreto-legge ho voluto però contestualizzare la gravità del problema, che coinvolge tutti noi e ho voluto chiarire le responsabilità di un Governo che, in oltre un anno, non ha saputo dare risposte al popolo italiano su un tema così importante.

onorevoli colleghi, l'Alitalia è la società aerea che porta le insegne del tricolore e che, grazie all'attuale nazionalizzazione, resta pur sempre la nostra compagnia di bandiera e continua quindi a interessare la politica italiana, nonostante le attuali vicende. Dopo la cessione in larga parte delle azioni ad Etihad, che ne aveva assunto la gestione nel 2014, è stato registrato il mancato ripristino di criteri di redditività, si è visto azzerare il patrimonio netto della compagnia tra il 2015 e il 2016 e si è adottato un ennesimo piano di ristrutturazione nel 2016. L'amministrazione straordinaria, come è stato più volte ricordato, si sta ora facendo carico di trovare delle offerte vincolanti per l'ottimizzazione degli *asset* del vettore aereo in questo senso, bisognerà capire come si articoleranno le nuove offerte e quale sia la più opportuna valorizzazione della compagnia: quindi il decreto-legge in esame è certamente funzionale allo scopo. La gestione commissariale, portata avanti da tre *manager* di assoluto valore, in questi ultimi anni ha operato per contenere i costi, incrementare l'efficienza, gestire meglio la liquidità e, soprattutto, mantenere i ricavi a livelli adeguati ad una così grande compagnia aerea. In tal senso va rammentato che, nell'epoca delle compagnie *low cost*, l'obiettivo di presidiare il mercato domestico con un prodotto che sia differenziato da quello dei voli a basso costo non è sicuramente un compito facile, ma non lo è nemmeno mantenere i collegamenti su rotte come quelle per il Medio Oriente o il Nord Africa, presidiate dalle grandi compagnie arabe, oppure sulle rotte europee, contro dei colossi come Lufthansa e Air France-KLM, ovvero sulla rotta verso la Russia, presidiata dalla compagnia di bandiera russa Aeroflot. Quello che va apprezzato è quindi ora lo sforzo per razionalizzare le rotte esistenti e per incrementare l'efficienza nell'utilizzo della flotta. Sono tutte azioni che hanno consentito anche una piccola crescita dei ricavi, che però rappresenta a mio avviso un'importante inversione di tendenza. Al contempo registriamo un'azione positiva dei commissari straordinari per contenere i costi attraverso una revisione e un'ottimizzazione della struttura organizzativa, l'internazionalizzazione di diversi servizi di bordo, la rinegoziazione dei contratti esistenti con i fornitori, il ritorno alla gestione diretta delle attività di cargo. Diversi passi avanti sono stati fatti anche sul piano delle relazioni industriali, anche se va ricordato

Grazie a questi strumenti è possibile gestire quasi 1.500 figure professionali, di volo e di terra, che altrimenti graverebbero interamente sull'azienda. Evidenziati gli aspetti comunque positivi di una gestione commissariale certamente non facile, va detto che uno dei principali indicatori di *performance* non è positivo: Alitalia perde mediamente passeggeri (anche se ne guadagna sul lungo raggio, cioè sulle rotte più redditizie), tiene su ricavi (come detto addirittura aumentandoli nel primo trimestre di quest'anno, rispetto al primo trimestre dello scorso anno) ma soprattutto riesce a ridurre le perdite operative nell'ultimo anno rispetto al precedente.

Al contempo, bisogna tenere conto dei limiti posti alla conferma del prestito all'Alitalia, che potrebbe costituire aiuto di Stato, ove rinnovato e non restituito. poi la solita domanda, che insegue l'Alitalia e la storia della sua cessione: può un Paese a larga vocazione turistica come l'Italia non possedere un vettore aereo di bandiera? Anzi: può un Paese come l'Italia rinunciare alla propria compagnia aerea? Bisogna cioè chiedersi se vale la pena cedere un *asset* strategico per il nostro Paese, come quello del trasporto aereo, in un momento in cui l'apporto al PIL dato dal turismo fiorisce e l'economia del trasporto aereo ha potenzialità e numeri di crescita molto importanti. Tutto sommato, ritengo che la storia dell'Alitalia non sia poi così diversa dalla storia del Paese Italia, per le tribolazioni e per il rapporto con gli altri Paesi. E, come per il Paese Italia cerchiamo una via per farci rispettare, così anche per l'azienda Alitalia - che a me piace sempre e comunque definire compagnia di bandiera dobbiamo trovare il sistema ideale per andare avanti nella maniera migliore per non disperdere un patrimonio così importante. La soluzione? Secondo me ha un nome: *confidence*; anzi, lo traduco in italiano: la fiducia. Grazie alla fiducia che in quest'ultimo periodo gli utenti stanno ritrovando, i ricavi nel primo trimestre del 2018 sono aumentati del 6 per cento (lo ricordo anch'io) e le perdite operative si sono dimezzate. Stefano Paleari, uno dei commissari straordinari - peraltro mio concittadino - lo ha indicato nel corso dell'audizione alla Commissione speciale del Senato. Parlando dei ricavi in termini concreti, questi si attestano a 597 milioni di euro, con una crescita del 4 in cui i ricavi da passeggeri crescono del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2017. E l'EBITDA, esclusi i ricavi e i costi non ricorrenti, riduce il rosso di 111 milioni di euro (nel periodo peggiore dell'anno per le compagnie). Lo stesso più o meno dicasi per il risultato operativo. Non dobbiamo dimenticare anche, come ha sottolineato il presidente dell'ENAC Riggio, che il perdurare della crisi dell'Alitalia potrebbe comportare grandi difficoltà anche sull'aeroporto di Fiumicino, principale scalo italiano della compagnia. Per concludere, oggi siamo chiamati a una scelta politica necessaria e urgente, per consentire alla nostra compagnia e a chi l'amministra di non dover volare a vista, ma di poter progettare e operare rispetto a un orizzonte temporale almeno di medio periodo.

Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, la scelta dei commissari da parte del Ministero dello sviluppo economico poco più di un anno fa per la gestione dell'amministrazione straordinaria dell'Alitalia che, come sappiamo, prevedeva centottanta giorni di tempo per presentare un piano di risanamento della compagnia, alla luce dei fatti, non si è rivelata propriamente consona alla problematica della compagnia aerea stessa. Il settore delle compagnie aeree è un *business* complesso e dalle mille variabili, che richiede competenze specifiche, come ha evidenziato il professor Intrieri, stimato esperto del settore aeronautico, nel suo intervento in Commissione speciale le scorse settimane. Intrieri, inoltre, ha evidenziato che nessuno degli amministratori delegati dell'Alitalia degli ultimi vent'anni proveniva dal settore aereo, il che è un caso unico al mondo. Nel caso in specie, per la gestione commissariale si è pensato ad ingaggiare sì un esperto, il professor Paleari, con ampissima esperienza in campo accademico, ma che forse non ha trovato il giusto coordinamento con la triade commissariale per disegnare una strategia avvincente. Il commissario Gubitosi, per sua stessa ammissione in recente audizione, è alla sua prima esperienza. Per quanto riguarda il commissario Laghi, non può passare inosservato il fatto che il conferimento dell'incarico commissariale era il suo ventiquattresimo incarico contemporaneo: quindi una situazione così grave e complessa, come quella del nostro vettore nazionale, che richiedeva tutta l'attenzione, si è vista probabilmente penalizzata dai numerosi impegni del commissario. La nomina dello stesso Laghi, altresì, è stata oggetto di un esposto all'Anac da parte del nostro Gruppo parlamentare, in quanto presentava profili di illegittimità, non rispettando praticamente nessuno dei requisiti relativi alle nomine dei commissari impartite dal decreto ministeriale L'Anac, con delibera n. 699 del 28 giugno 2017, ci ha dato ragione, dichiarando legittime le perplessità di chi sosteneva la possibile esistenza di un conflitto di interessi da parte di Laghi, in quanto pareva difficile che, avendo ricoperto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione di Midco SpA (la nuova società creata da CAI nel momento dell'ingresso di Etihad nell'azionariato Alitalia), non avesse mai partecipato all'amministrazione che ha portato Alitalia nelle condizioni attuali, cioè pessime.

i commissari, che in quel momento avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso della vendita, si sono invece limitati a effettuare una perizia interna che ha trovato congruo il prezzo. I dati oggettivi, però, erano altri e andavano approfonditi, tenuto conto della situazione contabile della compagnia. Quello di Heathrow è uno degli aeroporti europei in cui la fascia aerea si paga a caro prezzo ed è forse l'unico aeroporto al mondo dove si possono comprare e vendere diritti di atterraggio e decollo come se fossero titoli di borsa. Difficile quindi effettuare una perizia attendibile. Ma considerato che solo due anni prima la stessa Alitalia aveva venduto uno *slot* alla Continental per 30 milioni di euro, bastava farsi due conti e a quel punto sì che si potevano incassare dalla vendita a Etihad oltre i 60 milioni di Contestualmente alla vendita, Alitalia concordava il pagamento di un affitto piuttosto alto all'acquirente per il diritto di decollo e atterraggio dai medesimi slot di 3,5 milioni l'anno con un vincolo quinquennale. È evidente che i commissari avrebbero dovuto fare altri approfondimenti, visto che tutta questa trattativa ha penalizzato pesantemente Alitalia e ha presumibilmente contribuito al suo fallimento. In conclusione, proprio prendendo spunto dalle difficoltà di gestione e amministrazione della compagnia aerea non colte sin da subito dai commissari, si rileva la necessità che il Parlamento possa intervenire con maggiore incisività nelle vicende dell'Alitalia e di ogni altro *asset* strategico per il nostro Paese, e pertanto si concorda con una proroga nel corso della quale chiedere maggiore trasparenza, con la pubblicazione dei dati economici e tecnico-amministrativi con cadenza prefissata, affinché chiunque possa anche esercitare in ogni momento il monitoraggio della situazione.

quella che era una semplice proroga del finanziamento ponte è diventata un'analisi approfondita da parte di questo nuovo Parlamento, che non so quanto durerà, ma che almeno ha avuto modo di discutere e approfondire Ebbene, al di là dell'esame del decreto-legge, la Commissione speciale della quale mi onoro di far parte - che è stata, almeno in questo caso, un'esperienza importante per quanto mi riguarda, essendo io alla prima legislatura

agli esperti del sistema aeroportuale e degli aerotrasporti. Insomma, si è cercato non solo di dare un senso un senso a una proroga, ma di capire quello che si voleva fare di questa compagnia, quello che era questa compagnia e come se si fosse arrivati all'epilogo di un prestito ponte, quindi al commissariamento dell'azienda e, di conseguenza, alle scelte che si sono fatte nel tempo.

si sono cambiati dai sette ai nove amministratori delegati, nessuno dei quali si è mai occupato di aviolinee e compagnie

siete andati in quella direzione? Ebbene, qualcuno molto più autorevole diceva in quest'Aula: che a pensar male si fa peccato ma di solito si indovina. Da quando è entrato il socio (senza far nomi: Etihad) abbiamo assistito a un depauperamento della compagnia, quasi con l'obiettivo preciso e specifico di mangiarsi la compagnia, puntando, in un momento storico in cui si stava lanciando l'alta velocità (quindi, la ferrovia), sul domestico e annientando quasi il lungo raggio, andando a fare quelle operazioni, come qualcuno prima ha ricordato, della vendita degli *slot* in un aeroporto fondamentale come, per esempio, quello vendendo - così ci hanno riferito in Commissione - *slot* che avevano un valore dai 70 agli 80 milioni di euro a poco più di dieci milioni di euro, con un danno enorme per la compagnia. Ma non basta questo: non basta. Il conto economico, l'ultimo sul quale abbiamo potuto discutere, evidenzia che, in particolare per quanto riguarda i *leasing* degli aeromobili a lungo raggio,

un punto di eccellenza per la manutenzione e la sistemazione di motori, dove tutto il mondo veniva ad imparare. Oggi, quegli stessi ingegneri sono fuori a lavorare per le altre compagnie.

Non vogliamo parlare poi dei derivati e di tutto il resto, ma voglio che i colleghi riflettano su un argomento. Possiamo noi affidare a un nostro concorrente i nostri interessi? Ma voi, singolarmente o strutturati in azienda, affidereste mai ai vostri concorrenti i vostri interessi? È una follia. Una follia! Un'altra

come mai tutti questi applausi e sostegno per Air Italy, quando la nostra compagnia di bandiera, come ricordava prima il senatore Caliendo, ha un marchio riconosciuto nel mondo (come la Ferrari del resto), con un grande valore per la qualità (in ogni caso siamo valutati ancora come come una compagnia di bandiera di grandissimo livello). Come mai, con un marchio di questo tipo, con i capitani coraggiosi che l'avevano costituita, con la voglia di andare avanti, con la necessità di mantenere aperta un'azienda di questo genere, facciamo l'applauso e sosteniamo Air Italy? Io qui non so chi mi potrà rispondere: credo nessuno. In ogni caso, è la questione che ci siamo trovati di fronte. Pensate: ci hanno chiesto di parlare del prolungamento del prestito ponte e ci siamo trovati di fronte a questo disastro. Da questo punto di vista, però, c'è da dire che l'attività commissariale ha svolto un lavoro importante e che, se oggi siamo qui a discutere di questo con una prospettiva, dobbiamo ringraziare la gestione commissariale. Chiudo su una questione. Trovo fuori luogo e anacronistico che l'unico mandato dato ai commissari sia quello per la vendita dell'azienda. *(Applausi del senatore Dal

Si diceva come questo decreto-legge detti le misure per cercare di assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali che fanno capo all'Italia. Ricordo anche io come differisca al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento di tali procedure e prevede, inoltre, la proroga al 15 dicembre 2018 del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, come originariamente previsto dal precedente

come già dal 2008 il Parlamento e la politica italiana si siano impegnati per cercare di salvare questa importante azienda.

Per quanto riguarda il lavoro della Commissione, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a importanti audizioni rappresentanti sindacali di tutte le sigle, che non sto qui a citare. Tutti gli attori si sono presentati, incluso il collegio commissariale della procedura. Abbiamo audito anche l'ENAC, e il comitato di sorveglianza nella procedura di amministrazione straordinaria, che hanno permesso di aggiornare un quadro importante e preoccupante. preoccupazioni erano soprattutto riguardanti il personale. Sono stati fatti dei tagli importanti, ma soprattutto i sindacati hanno espresso

Per quanto riguarda la politica industriale abbiamo potuto rilevare delle criticità, legate ad esempio esempio alla riduzione dei voli a lungo raggio e ci è stato spiegato come effettivamente questo rappresenti

una relazione contenente una serie di punti dettagliati; tuttavia, se questo può servire a mantenere un contatto ancora più stretto con la parte politica, ben venga. In conclusione rilevo che il nostro Gruppo ha seguito

si sia creato un clima di fiducia, che forse è anche l'elemento che ha consentito, durante questa fase di commissariamento, di ridare slancio ad Alitalia. Finalmente sembra ci sia l'opportunità di provare a guardare il futuro, forse anche con qualche possibilità in più di ampliare l'orizzonte delle prospettive. La ripresa della compagnia aerea a partire dal maggio 2017 (ricordiamo che questa è la data di avvio dell'amministrazione straordinaria) risulta essere abbastanza sostenuta; abbiamo visto i dati, che sono pubblici, e sappiamo anche da dove stavamo partendo. I buoni risultati raggiunti sembrano dovuti in particolare proprio a una ritrovata fiducia della clientela rispetto alle sorti della compagnia ciò ha reso possibile un aumento dei ricavi, connesso essenzialmente all'incremento del numero dei passeggeri. Questo è un punto da tenere sicuramente in considerazione, perché poi si registra una crescita stimata per il primo semestre del 2018, 2018, con un aumento dei ricavi del 4-5 per cento e un incremento in particolare proprio dei passeggeri sui voli intercontinentali. Le azioni della gestione commissariale, come veniva ricordato prima, hanno consentito quasi una sorta di programmazione per i prossimi mesi.

risorse in misura sufficiente a garantire la compagnia in un'azione di medio termine, primo elemento necessario - e lo ribadisco ancora una volta per recuperare fiducia e garantire agli utenti e a chi si serve di Alitalia di poter avere uno sguardo anche positivo. Quindi fiducia. Fiducia, però, che non deve soffermarsi solo sul presente. Abbiamo bisogno di guardare al futuro, abbiamo bisogno di avere uno slancio ulteriore per provare a rafforzare ulteriormente il posizionamento strategico della compagnia aerea. Quali interventi sono necessari? Anche in questo caso li abbiamo ascoltati e noi, come Partito Democratico, abbiamo provato anche a ribadirli:

ha una posizione dominante: circa 200 movimenti al giorno, una quota di mercato del 65 per cento, una grande quantità di *slot*. Dobbiamo guardare con molta attenzione a questo *asset* perché da esso possono partire opportunità anche per il Paese e lo dico anche da milanese, non solo da lombarda. Linate è un aeroporto molto amato dai milanesi che lo vedono come collegamento diretto alla città. Sappiamo anche che esiste un progetto che riguarda una fermata della metropolitana proprio a Linate, che garantirà un ulteriore collegamento e una vicinanza ulteriore

non di riduzioni. Stiamo parlando di sinergie tra forze che stanno svolgendo con professionalità i loro compiti. Linate è anche il City Airport migliore d'Europa. Offre 20 destinazioni. Possono crescere facilmente senza modificare l'attuale numero di passeggeri in transito. Siamo convinti, proprio per questo, che Linate sia un aeroporto strategico per lo sviluppo e il potenziamento di Alitalia in termini di ricavi, fatturato e voli.

vorrei utilizzare nella mia riflessione. Per non svendere c'è bisogno di tempo, ma i tempi devono essere certi e la politica deve assumersi la responsabilità di tempi certi per portare a compimento anche i progetti di accompagnamento già avviati. Sappiamo benissimo quali sono le scadenze. Gli incarichi assegnati ai commissari sono prossimi alla scadenza. Entro il 31 ottobre 2018 devono essere concluse le procedure di gara per la cessione dei complessi aziendali. Entro il 15 dicembre il prestito concesso alla compagnia aerea deve essere restituito. Pertanto, è possibile rinunciare alle opportunità, è possibile rinunciare

proseguire, sempre con data certa, in un percorso che ha già dato dei risultati. La mancata decisione sul futuro di Alitalia nei prossimi mesi, oltre a generare vantaggi competitivi in favore di altre compagnie aeree,

che possano garantire davvero la continuità operativa di Alitalia nei termini che abbiamo provato prima a descrivere. Forse sarebbe tempo - concedetemelo - che la politica si assumesse, anche in questa circostanza, una responsabilità maggiore; intendo con politica non solo chi aveva i numeri nella scorsa legislatura, ma anche chi questi numeri

Passando alla disamina del provvedimento, bisogna ricordare che il decreto‑legge in esame mette in atto una serie di misure urgenti per assicurare il completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia. In particolare, sposta al 31 ottobre 2018 il termine per l'espletamento di tali procedure, previste dal decreto-legge n. 148 del 2017, e proroga fino alla fine di quest'anno la durata del finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, già disposto dal decreto-legge n. 50 del 2017, che è poi stato incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, sopprimendo contemporaneamente le disposizioni che ne prevedevano la restituzione entro il termine dell'esercizio finanziario. Tutto questo, evidentemente, per dare un certo respiro e beneficio alla difficile situazione economica della società. Alitalia Alitalia è stata ed è ancora oggi la nostra compagnia aerea di bandiera; ricordo che ha iniziato le sue operazioni di volo nell'immediato dopoguerra, esattamente nel 1947. la situazione attuale della Società Aerea Italiana (SAI), che è in amministrazione straordinaria, ricordo che essa ha avviato le operazioni il 1° gennaio 2015, dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI, che detiene in Alitalia una quota di controllo pari al 51 per cento. Il 49 per cento delle azioni è di proprietà di Etihad Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Fallito il piano di rilancio di Etihad, che prevedeva il *break even* (il punto di pareggio tra le entrate e le uscite) nel 2017, la compagnia, che non ha un bilancio positivo ben dal 2009, ha subìto perdite per 500 milioni di euro Poi, nell'aprile del 2017, ha siglato un preaccordo sui tagli e indetto un *referendum* tra gli allora 12.500 dipendenti. Il 24 aprile 2017 i lavoratori di Alitalia hanno, però, bocciato il preaccordo, che prevedeva una ricapitalizzazione in cambio di in cambio di tagli al personale, aprendo così la strada al commissariamento della compagnia e, in mancanza di nuovi finanziatori, alla dichiarazione di insolvenza da parte del tribunale. Il 2 maggio 2017 il Ministero per lo sviluppo economico ha nominato i tre commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari per occuparsi dell'amministrazione straordinaria della società. Per garantire l'operatività nei mesi immediatamente successivi al commissariamento, il Governo ha concesso un prestito ponte di oltre 600 milioni. L'evoluzione della situazione di Alitalia nel corso

accadendo ora, se non la rifinanziamo) e per due volte rinata nell'arco di dieci anni. Oggi noi, con questo decreto di finanziamento, dovremmo contribuire a farla rinascere per la terza volta, il tutto, chiaramente, con i soldi dei cittadini italiani. Questo credo che sia un motivo di riflessione, perché per l'araba fenice, come sappiamo tutti, risorgeva dalle proprie ceneri, mentre Alitalia risorge con i soldi dei contribuenti di questo Paese. Negli ultimi anni, imprenditori, banchieri e *manager*, con il decisivo contributo delle casse pubbliche, si sono esibiti spesso in una sorta di gioco di prestigio finanziario pur di evitare il *crack* della compagnia aerea, che ha smarrito da tempo immemorabile la rotta dei profitti. Eppure, quanto è successo nelle ultime settimane, e quanto ancora avviene in questi giorni tra polemiche politiche e scaricabarile assortiti, sembra davvero l'ultima possibilità per vincere una partita che a molti sembra dall'esito già irrimediabilmente compromesso per la terza volta. Un po' di storia. La società opera sia nel settore passeggeri che in quello cargo. Dal novembre 2014 al 2 maggio 2017 il presidente della compagnia è stato Luca Cordero di Montezemolo, e devo dire che il presidente Montezemolo, visti i risultati e le perdite di quegli anni, sicuramente non verrà ricordato molto positivamente nei libri di storia delle prossime generazioni. Le prime peripezie industriali e finanziarie prendono le mosse negli anni Novanta, quando, a fronte delle prime, evidenti difficoltà economiche, l'allora *premier* Romano Prodi lancia la prima privatizzazione. Siamo nel 1996 e la quotazione in borsa del 37 per cento della società non porta i frutti sperati. Un secondo tentativo verrà poi fatto nel 2006, sempre da Prodi, con una modalità questa volta diversa: invece della borsa, si sceglie di mettere sul mercato un altro 39 per cento con una procedura di gara che però fallisce fin da subito, perché chi vi doveva partecipare, non appena va a vedere i conti della società, prende paura talmente erano in rosso. Siamo ancora Siamo ancora negli anni Novanta quando si prova a mettere in campo una prima alleanza strategica con il vettore KLM. La *partnership* però fallisce e la compagnia olandese decide nel 2000 di ritirarsi subito dall'operazione in maniera unilaterale.

scende in campo la Compagnia aerea italiana (CAI), una cordata guidata allora da Roberto Colaninno e da altri investitori come Benetton, Riva, Ligresti, Marcegaglia e Caltagirone. Alla cordata partecipa anche una banca di peso come Intesa San Paolo, allora guidata da Corrado Passera. La parte sana della compagnia viene rilevata dalla CAI per 300 milioni mentre tutto il passivo, ovvero circa 2 miliardi di euro, viene messo in una *bad bank* e diventa debito di Stato, quindi a carico di tutti i cittadini di questo Paese. Nel mese di marzo 2017 Alitalia è di nuovo sull'orlo del fallimento: si prevede che la cassa disponibile, nel giro di un mese, non sia sufficiente né per il rifornimento dei velivoli né per pagare gli stipendi.

Arriviamo ad oggi: compito dei commissari straordinari è di individuare l'offerta migliore, per poi aprire la fase della negoziazione in esclusiva, per entrare nel dettaglio di alcuni nodi fondamentali,

- è lo scopo dell'amministrazione straordinaria, e che per questo si presta a varie considerazioni sulla gestione commissariale. La prima considerazione è che la gestione corrente - l'abbiamo visto in Commissione dopo aver audito i tre commissari - è stata comunque positiva, con significativi miglioramenti dei conti. Non si cada però subito nell'illusione, nell'inganno di pensare che Alitalia sia rinata, perché assolutamente non lo è. Nel primo trimestre ha perso due milioni di euro al giorno. È vero che si tratta della stagione meno redditizia dell'anno, tuttavia questa cifra ci fa pensare ai tempi più bui. A favore del lavoro dei commissari va detto e sottolineato che gli stessi numeri del trimestre dicono anche che, rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti, sono aumentati i ricavi e sono calate significativamente le spese e questo di fatto promuove la gestione ordinaria. Concludendo, credo sia assolutamente prioritario che quanto prima si ponga termine alla gestione commissariale e si proceda alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione con degli obiettivi e strategie adeguati soprattutto alla nuova richiesta di mobilità globale. Questo chiaramente nell'interesse della società, nell'interesse dei lavoratori di Alitalia, nell'interesse dei lavoratori dell'indotto aeroportuale e nell'interesse dei cittadini Italiani, che fino ad oggi, grazie alle scelte degli ultimi Governi,

illustrato la posizione che abbiamo tenuto nella Commissione speciale, in questa fase un po' particolare dei lavori del Parlamento, in cui però l'eterna questione dell'Alitalia ha trovato modo di spuntare. Parlo di eterna questione perché è molto tempo che il Paese si misura con la vicenda della compagnia che un tempo avremmo definito di bandiera e quindi siamo preoccupati di quella che può essere la prospettiva. non sappiamo quali sorti toccheranno all'Italia in termini di Governo, ma certamente della questione ci si dovrà occupare. Non vorremmo che la concitata fase politica potesse cagionare danni alla gestione e alle prospettive dell'Alitalia, il cui valore occupazionale e strategico e la cui ricaduta sul turismo hanno l'importanza che tutti abbiamo sottolineato. Il nostro Gruppo, voterà a favore della conversione di questo decreto-legge perché ritiene che le misure già discusse e illustrate siano indispensabili. Vogliamo però cogliere l'occasione di questo dibattito per far presente a chi avrà responsabilità di governo nella media prospettiva - in queste ore è un'incognita assoluta e quindi parliamo veramente in totale buona fede e ignorando le prospettive questo dibattito ha messo in luce gli errori commessi anche in fasi che sono state vantate come fantasmagoriche: la vicenda Etihad, gli esponenti preclari del mondo industriale che avevano prospettato questa soluzione come una soluzione mirabolante. Ci sono addirittura aspetti inquietanti di questa vicenda che dovranno essere approfonditi, forse più nelle sedi giudiziarie che altrove. Nella storia passata di Alitalia ci sono pagine di sprechi e costi eccessivi e anche pagine che hanno dimostrato come il mondo imprenditoriale (che spesso dà lezioni a quello politico) chiamato a gestire questa vicenda, poi non ne fu capace. l'operato dei Governi di centrodestra, chiamati a difendere la funzione strategica di Alitalia, allora sì, non vendendola ai francesi e mantenendo la struttura sotto controllo italiano per evitare di perdere scali italiani, anche quelli di grande rilevanza turistica (praticamente tutti, perché l'Italia è tutta visitabile e meta ambita

che è forse difficile immaginare un futuro roseo, in autonomia e in solitudine, perché i macronumeri sono impietosi. Basta vedere la grandezza delle compagnie aree, che ci hanno ricordato i commissari intervenuti in audizione presso la Commissione speciale

prima o poi avrà un Governo.

recante misure urgenti per la situazione attuale della compagnia di bandiera, per la quale si prevede una proroga del prestito di 900 milioni di euro e il processo di vendita. Abbiamo richiesto delle audizioni formali, che sono risultate davvero importanti sia dal punto di vista della trasparenza sia dal punto di vista dell'attività parlamentare. Durante l'esame in Commissione speciale abbiamo molto apprezzato gli interventi, indistintamente, di tutti i colleghi senatori. La problematica inerente ad Alitalia ha quindi avuto una grande rilevanza, da parte di tutti i Gruppi parlamentari, sottolineando che, in un Paese come il nostro, Alitalia è un *asset* strategico. Ciò risulta evidente per una nazione come la nostra, a forte vocazione turistica, con un mercato manifatturiero che è tra i primi in Europa, e per un territorio pieno di ricchezze culturali, bellezze geografiche e storiche, in cui il mercato del trasporto aereo - si tratta di un dato tra il secondo e il terzo posto in Europa e al sesto posto nel mondo. Come Gruppo parlamentare abbiamo approfondito al massimo la tematica, studiando a fondo la poca documentazione amministrativa e tecnica che era stata messa a disposizione, anche dai commissari, prima delle audizioni. Abbiamo riportato alla luce voci di ingenti costi fissi non ancora chiariti ed abbiamo anche cercato di capire dove possono essere le perdite attuali di Alitalia, che paradossalmente risulta essere l'unica compagnia aerea d'Europa in perdita, in un mercato che da

economica inerente alla gestione di Etihad e anche a quella commissariale. Apprendiamo da fonti di stampa che fin da subito sono stati rilevati dati non chiari, soprattutto nei primi tre mesi del 2017, quando l'azienda perdeva diversi milioni di euro. È venuto a galla, grazie anche alla nostra insistenza in audizione, che sono stati venduti degli *slot* di alto valore ad un prezzo che potrebbe essere non congruo, quindi recando ulteriore danno alla compagnia e che risultano

Abbiamo rilevato anche dei problemi riguardo al *wet leasing*, ovvero riguardo al noleggio degli aeroplani. Ci sono diverse società di cui non si conosce la provenienza, ci sono società in Irlanda e società che fanno capo all'Italia, ma il problema è quanto costa il *wet leasing* ad Alitalia. In seguito alle audizioni, il commissario Laghi ha fatto sapere a mezzo stampa e non in audizione che esistono crediti da recuperare da Etihad pari a circa 600 milioni è quindi evidente che il nostro emendamento in Commissione speciale sia giustificato dalla possibilità di implementare un controllo diretto e anche proattivo sull'operato dei commissari e sulla precedente gestione. La proroga del prestito non può essere vanificata e deve essere fortemente limitato il rischio di perdita ulteriore di soldi statali, quando invece questa proroga deve avere lo scopo di salvaguardare Alitalia, i suoi dipendenti e tutto l'indotto, che spesso non viene citato. Proprio in virtù di un vero cambio di rotta - per rimanere in tema - non si può più andare avanti sulle strade già percorse, ma bisogna finalmente risolvere anche questa annosa vicenda, che ormai, a cadenza di due o o tre anni, comporta mattanze sociali, perdite economiche per il Paese a vantaggio di altri e ulteriore cassa integrazione, nonché disoccupazione e questa è una sconfitta per un Governo. Il mercato aereo in Italia è stato aggredito in modo incontrollato e anche disinteressato da parte dei vari Governi. È stato concesso di tutto a chi, di fatto, ha ha aumentato la precarietà e ridotto i minimi salariali, in alcuni casi non pagando nemmeno una tassazione equa nel nostro Paese, ma facendo ciò che voleva. La politica ha quindi fatto la sua parte fino ad oggi, già, ma andando contro gli interessi dell'Italia stessa, compartecipando alla distruzione dei nostri *asset* a beneficio di terzi, includendo l'opera ingannevole di posizionare *manager* presentati come grandi esperti, ma che di fatto hanno palesemente dimostrato di saper fare interessi ben diversi da quelli delle aziende che avevano avuto l'onore di gestire. Le verità vengono fuori giorno dopo giorno, inesorabilmente, anche grazie a chi dedica tantissimo tempo alle tematiche specifiche, approfondendo a favore di chi ha sempre subito ingiustamente, come i dipendenti e i cittadini italiani, che sono stati male informati, sempre per far ricadere le colpe su chi di fatto non ne ha avute. Bene dunque la proroga del prestito, fatto più che responsabile ai fini della continuità della compagnia di bandiera; ma non possiamo pensare di lasciare che la vicenda Alitalia solchi ancora il percorso di sempre, nel silenzio-assenso. L'attività parlamentare deve tornare ad essere attiva nelle vicende importanti del Paese. Riteniamo più che opportuno aiutare il nostro *asset* strategico a recuperare crediti, invece di fare debiti ulteriori, perché ad oggi non ci risultano utili. Nonostante il potere dei commissari rispetto alla risoluzione di contratti sfavorevoli alle casse aziendali, nonostante anche il cattivo operato della precedente amministrazione e di quella che c'era ancora prima dei capitani coraggiosi, c'è assoluta necessità dunque di approfondire in modo trasparente. La procura farà altrettanto il suo percorso, ma anche noi parlamentari siamo assolutamente chiamati a fare il nostro lavoro.

Signor Presidente, onorevoli senatori colleghi, il mio intervento questa sera è per ricordare che oggi è il sesto anniversario del sisma che ha colpito nel 2012 il territorio della mia Regione, l'Emilia-Romagna,

i 300 feriti, le 45.000 persone sfollate e i danni inerenti che hanno investito i territori delle Province di Modena, Ferrara, Bologna e Reggio Emilia. Nel corso di questi anni, grazie allo spirito di collaborazione che ha visto coinvolti cittadini, imprese, professionisti, associazioni, volontari, dipendenti pubblici e istituzioni, l'Emilia-Romagna non si è mai fermata. Sono stati fatti grandi passi in avanti nel percorso della ricostruzione: ben l'87 per cento delle ricostruzioni, che presenta comunque aspetti e questioni ancora da risolvere. A sei anni di distanza l'area del cratere, nonostante gli eventi sismici, continua a crescere e a produrre grazie a fabbriche, a capannoni e a strutture nuove rese più sicure ed efficienti. Oltre 10.000 attività economiche, negozi, uffici, botteghe artigiane ed oltre 3.000 strutture produttive industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi hanno ottenuto, grazie anche all'impegno del commissario delegato dal Governo (il presidente della Regione Stefano Bonaccini) e al lavoro congiunto dei parlamentari (deputati

cento delle 16.500 costrette a uscire nel 2012 dopo le scosse, e quasi 14.000 le abitazioni rese di nuovo agibili. Il Governo Gentiloni Silveri, in continuità con i Governi di centrosinistra precedenti, con la legge di bilancio per il 2018 ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per le popolazioni e i territori colpiti Voglio ricordare le misure contenute nella finanziaria: prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU; prorogata al 2019 la possibilità per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici, di sospendere gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; incrementato di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020